apre una nuova finestra"). Onorevoli Colleghi, comunico che il Presidente del Senato ha ricevuto la seguente lettera del Presidente del Consiglio dei ministri: «Roma 21 febbraio 2007 Onorevole Presidente, La informo che in data odierna, tenuto conto del voto espresso dal Senato della Repubblica, ho rassegnato al Capo dello Stato le dimissioni del Gabinetto da me presieduto. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha invitato il Governo a restare in carica per il disbrigo degli affari correnti. *f.to* Romano Prodi». Con le dimissioni del Governo l'attività del Senato, legislativa, di controllo e di indirizzo, viene sospesa in coerenza con i princìpi generali dell'ordinamento costituzionale, che considera il Governo interlocutore indispensabile del Parlamento. Di conseguenza, dopo l'annuncio delle dimissioni, l'Assemblea e le Commissioni possono essere convocate limitatamente allo svolgimento di attività legislative correlate a scadenze costituzionali (quali i decreti-legge) o per adempimenti inerenti ad *interna corporis* (quali autorizzazioni a procedere in giudizio, questioni di insindacabilità, bilancio interno). Le Commissioni sono inoltre autorizzate a esprimere il proprio parere su atti del Governo nonché a proseguire le procedure informative già avviate, avendo cura di evitare richieste incompatibili con la posizione del Governo dimissionario. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha preso atto del calendario che, in relazione alla crisi di Governo in corso e a quanto previsto dall'articolo 55, comma 6, del Regolamento, prevede l'esame dei soli decreti-legge in scadenza. Pertanto, questa mattina riprenderà la discussione del decreto-legge di recepimento di direttive comunitarie. Nella seduta antimeridiana di giovedì 1° marzo inizierà, ove concluso dalle Commissioni competenti, l'esame del decreto-legge sulla prevenzione della violenza nelle competizioni calcistiche, che proseguirà la settimana successiva.

e per l’adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all’assistenza a terra negli aeroporti, all’Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio,

a me sembra che oggi debba prevalere la valutazione politica sulle esigenze istituzionali. Noi capiamo la difficoltà odierna - c'è un decreto in scadenza - ma riteniamo che i lavori dell'Assemblea, così come abbiamo detto nella Conferenza dei Capigruppo che si è appena svolta, debbano essere sospesi in assenza di un Governo e per la confusione che oggi caratterizza

Presidente, non siamo insensibili al fatto che c'è un decreto, che ci sono esigenze, che la Costituzione prevede comunque che, anche a Camere sciolte, si debba tenere seduta per l'esame dei decreti, tuttavia, la confusione oggi è tale che non permette all'Assemblea di proseguire i lavori e pertanto chiedo che siano sospesi.

noi ci siamo espressi in maniera leggermente difforme, ma per un motivo meramente istituzionale, nel senso che siamo costretti, credo da un punto di vista costituzionale-regolamentare, a riconoscere la facoltà della maggioranza - nel caso lo voglia - di portare avanti l'esame dei decreti-legge, perché questo è previsto

Si tratta di stabilire cosa fare rispetto a queste due esigenze diverse: da un lato, il riconoscimento - perché è nei fatti - della facoltà di poter, appunto,

di crisi di Governo, però abbiamo voluto privilegiare e privilegiamo l'aspetto politico. Noi riteniamo che non si possa procedere di fronte ad una situazione complessa,

forse potrebbe anche essere probabile, riteniamo di privilegiare questo aspetto politico. Pertanto, abbiamo espresso e confermiamo la nostra contrarietà al calendario e invitiamo a non procedere nelle attività di Aula fin quando non si chiarirà la

Presidente, credo che su una questione lei farà piena luce, è cioè che non c'è un problema di calendario. Questo chiarirà un primo punto, ma penso che lo farà lei compiutamente e quindi non mi diffondo sulla questione. È la terza volta da ieri, Presidente, che affrontiamo questo argomento, che è già stato deciso, per ben due volte, dalla Presidenza dell'Assemblea, sia nella persona del presidente Marini che nella persona del presidente Calderoli e penso che toccherà a lei, per la terza volta, dire le stesse cose. Non accogliamo la richiesta dei colleghi dell'opposizione

che in queste circostanze il Parlamento possa - per quanto mi riguarda dovrei dire «debba» - esaminare i decreti.

che ci si possa riuscire e quindi, Presidente, chiedo di proseguire nell'andamento dei lavori già previsti dal calendario per la giornata di oggi. Signor Presidente, chiedo, con un richiamo al Regolamento, la possibilità di modificare l'ordine del giorno. Facendo riferimento all'articolo 56,

la situazione attuale ci dà e che, in questo caso, potremo soddisfare le richieste dei senatori che vogliono rimanere Sottosegretari. Annunciamo sin d'ora che daremo il nostro voto favorevole. Chiedo quindi di poter operare questo inserimento all'ordine del giorno. passiamo alle decisioni da assumere: innanzitutto - comincio dall'ultimo intervento del senatore Pirovano - non stiamo esaminando nessun calendario dei lavori. Le prerogative riservate dalla Costituzione e dal Regolamento al Presidente del Senato consentono, per sua libera scelta e decisione insindacabile, di mettere in discussione e di portare in Aula i decreti in scadenza.

non possiamo in alcun modo accettare le considerazioni o per meglio dire - cito testualmente - le esigenze politiche sopravanzate dai colleghi Casellati, Castelli e Tofani a fronte di prerogative costituzionali che Regolamento del Senato e Costituzione della Repubblica attribuiscono al Presidente del Senato. Ciò non è in alcun modo possibile né accettabile. È potere del Presidente, in base all'articolo 55, comma 6, del Regolamento, decidere di portare all'attenzione e alla discussione dell'Aula i decreti-legge in scadenza, nel merito del quale potere, cari colleghe e colleghi, non voglio sottolinearne, ma lo posso fare, il rilievo e l'importanza oltre che l'urgenza. Evidenzio che nel merito delle discussioni che stiamo facendo, cioè sulle modalità di voto, sulle procedure da assumere nella discussione e nelle votazioni di merito dei decreti, è naturalmente prerogativa dei singoli Gruppi, di maggioranza e di opposizione,

Mi spiace, senatore Castelli, ma questa è una prerogativa del Presidente, confermata da parte del Presidente nella Conferenza dei Capigruppo, ancorché, come correttamente è stato riferito, con l'opinione diversa di alcuni Capigruppo presenti, dell'opposizione o della minoranza, o quella che sino a questo momento è risultata tale. Così stanno le cose, senatore Castelli. Lei, come Capogruppo della Lega e altri colleghi, Presidenti dei Gruppi, avete ora tutte le possibilità e le prerogative che il Regolamento vi attribuisce e vi riserva per ostacolare il percorso del provvedimento *in itinere*. Signor Presidente, comprendo benissimo e condivido quanto lei ha detto. Però vi è un aspetto, a mio avviso,

far valere una valutazione di opportunità politica a fronte di una prerogativa di profilo costituzionale che penso tutti dobbiamo difendere. Nel merito, i Gruppi hanno poi la possibilità di utilizzare le norme regolamentari.

Senatrice Alberti Casellati, mi permetto ancora di insistere. Non si tratta di una modifica del calendario. Il calendario è rimasto esattamente lo stesso. Si fa riferimento esclusivamente a quei decreti‑legge, già all'attenzione delle Camere, in questo caso della nostra, che a norma di Costituzione possono essere esaminati dalle Camere medesime non solo in caso di crisi di Governo, ma anche - come lei sa - persino di scioglimento delle Camere.

è data facoltà ai singoli Gruppi di utilizzare le norme regolamentari per impedire od ostacolare il percorso o addirittura l'approvazione dei medesimi decreti.

il sistema complessivo delle banche e delle imprese italiane, per adeguarsi al nuovo regime di disciplina dell'adeguatezza di capitale delle banche, deve compiere uno sforzo, che ha destato preoccupazione anche in quest'Aula. Ciò mi porta a dire che l'Assemblea, in sostanza, riconosce l'urgenza di provvedere attraverso il recepimento delle direttive: proprio il fatto che è richiesto a banche e imprese uno sforzo per adeguarsi, significa che è opportuno che questo sforzo venga avviato il più presto possibile, considerando che comunque dovremo adeguarci.

manifestate circa l'adeguatezza organizzativa delle banche italiane, ovvero la struttura patrimoniale e organizzativa del sistema delle piccole imprese italiane. Prima procediamo, meglio è, da questo punto di vista.

In realtà, come è noto, tale requisito non è sempre rispettato, ma qui c'è un criterio di omogeneità che credo tutti riconoscano: esso non è per oggetto, ma è relativo alla necessità di adempiere ad alcuni obblighi comunitari

nel dicembre 2006); e, per la parte restante, in un'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione, quindi una decisione dell'Unione, che per essere utilizzata anche dal punto di vista finanziario, per rendere cioè utilizzabili delle risorse finanziarie nel nostro Paese, richiede la nascita della nuova Agenzia per i giovani.

su questo provvedimento. Data l'ampia illustrazione e la replica puntuale svolta dal senatore D'Amico, mi limiterò a toccare solo alcuni temi che giudico particolarmente rilevanti. Come è stato richiamato in discussione generale, si tratta di un provvedimento con un connotato prevalentemente tecnico, ma non per questo meno importante. La stessa necessità di rispettare degli obblighi comunitari incombenti che certamente ha ispirato questo provvedimento (è innegabile) non deve indurre a sottovalutarne la valenza positiva per l'economia e per il Paese. In particolare, vorrei riferirmi al cosiddetto accordo di Basilea 2: un accordo che, come è noto, è stato sottoscritto da tutti i principali Paesi. In Europa, in particolare, si è affermata la volontà davvero comune di pervenire ad una metodologia pienamente omogenea di valutazione del rischio e di allocazione del capitale e, di conseguenza, di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale delle banche e delle imprese di investimento. Con Basilea 2 credo che potremo garantire un'allocazione più razionale e più sofisticata del capitale delle nostre aziende di credito. Di conseguenza, si libereranno delle risorse finanziarie che il sistema bancario italiano potrà mettere a disposizione dei propri clienti, ovvero il sistema produttivo e le famiglie. Quindi, a mio avviso otterremo non solo un migliore grado di competitività del nostro sistema finanziario ma anche risorse finanziarie aggiuntive per il sistema delle imprese, anche per quelle di minori dimensioni, e per le famiglie. È vero, e credo che non possa essere disconosciuto, che l'*iter* di conversione di questo decreto-legge, che scade come sapete domenica 25 febbraio, ha in qualche misura forse limitato l'attività della Commissione prima e dell'Aula poi. In tal senso, anche se è un momento politico molto particolare, mi sento di fare mie le raccomandazioni del presidente Benvenuto e quindi di garantire in futuro che in Senato su provvedimenti di questo tipo (ve ne sono altri che prossimamente dovranno essere recepiti nel nostro ordinamento: mi riferisco ad esempio alla direttiva MIFID, alla direttiva sull'OPA) vi sia un calendario dei lavori pienamente adeguato, data l'importanza dei provvedimenti in questione.

e per l'adeguamento a decisioni, sempre in ambito comunitario, relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio. Pertanto, gli emendamenti 4.100, 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103,

x1.100 e x1.101 risultano improponibili in quanto estranei all'oggetto del decreto-legge. Risulta altresì improponibile l'emendamento x1.102, in quanto recante proroga di un termine già scaduto per l'esercizio di una delega

di una scadenza così indefinita sono assolutamente fuori luogo. Quindi abbiamo proposto di inserire scadenze assolutamente

Sarebbe lungo e doveroso discutere di quanto ha fatto o non ha fatto in passato la Banca d'Italia nell'adempimento dei propri doveri di controllo sul sistema bancario; lasciare tali oneri ancora aperti a variabili di questo tipo, e quindi a una sorta di facoltatività, ci sembrava altresì

Presidente, la presentazione di alcuni emendamenti da parte mia mi consente anche di svolgere qualche considerazione. Lei, molto correttamente, ha richiamato la prassi costituzionale (è un dato innegabile), ma siamo di fronte a questioni politiche di una certa rilevanza. Il relatore e la maggioranza hanno impedito anche la correzione di questioni tecnico‑formali assolutamente imprescindibili. Mi riferisco, in particolare, alla presenza nel titolo relative all'assistenza a terra negli aeroporti che è stato soppresso alla Camera dei deputati e che noi abbiamo il dovere di correggere, perché non possiamo approvare una legge con un titolo modificato dall'altro ramo del Parlamento, senza che possano intervenire modifiche. Ora, le preoccupazioni sorte

tutta la parte relativa a Basilea 2 all'interno di quel decreto perché possa essere data continuità di azione, riuscendo a salvaguardare eventuali rapporti giuridici insorti rispetto alla normativa secondaria approvata dalla Banca d'Italia sul finire del 2006, quindi senza pregiudicare assolutamente la parte normativa. Aggiungo che noi abbiamo presentato modestissime correzioni, che non sono state tenute in alcuna considerazione, anche di omogeneizzazione del testo perché abbiamo verificato terminologie diverse che prendono in esame la stessa materia. L'articolo 5 contiene un gentile *cadeau* al ministro Ferrero, ma come possiamo approvarlo in presenza di una crisi di Governo che investe l'intero Esecutivo? Quindi, invito la maggioranza a riflettere

che produce gli effetti auspicabili ricordati dal Sottosegretario. Per questi motivi, e senza entrare nel dettaglio tecnico di ciascun emendamento, sul quale mi sono soffermato in Commissione, do parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 1.

della disciplina finanziaria in Italia: è necessario e utile provvedere ad un riordino complessivo della normativa. Per questo è stato presentato a firma del relatore l'ordine del giorno G1.101 che indirizza il Governo

il Governo si conforma al parere del relatore per quanto riguarda gli emendamenti e circa gli ordini del giorno G1.100 e G1.101 esprime parere favorevole.

2, come sapete, è di estrema importanza, tanto che da due anni viene discusso nelle Aule parlamentari e nelle sedi tecniche, e coinvolge

non vi è stata neanche una piccola apertura nell'analisi dei nostri, ancorché minimi, cambiamenti, vale a dire nel contenimento delle spese che il sistema bancario dovrà addossare alle piccole e medie imprese per tutte le analisi tecniche, molto complicate, che tali imprese dovranno sostenere. Quindi, a nostro avviso, il metodo è assolutamente inaccettabile, così come non possiamo accettare

per rispondere alle osservazioni del collega, che dice che non stiamo lavorando in modo adeguatamente democratico e che dovremmo tenere conto di quello che è accaduto ieri, per suggerire ai colleghi di acquistare l'«Herald Tribune» di oggi: in prima pagina, c'è una grande fotografia, in cui tutti voi vi potete riconoscere mentre urlate e lanciate fogli di giornale. Dice la scritta: «Senatori italiani al lavoro». siamo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento, non mi pare che lei abbia aggiunto nulla da questo punto di vista.

delle preoccupazioni che venivano dal sistema delle piccole e medie imprese, in particolare per gli effetti derivanti dall'introduzione dell'accordo di Basilea 2, e degli effetti che si potevano riverberare, per così dire, sulle fonti di finanziamento. Con il senatore Cantoni abbiamo sollecitato la maggioranza e il rappresentante del Governo a tenere in considerazione che, nell'ambito dei poteri conferiti all'Autorità di vigilanza, rispetto alle informative che le banche debbono rendere al pubblico sugli aspetti rilevanti per la vigilanza di stabilità fosse inserito anche il livello delle riserve tecniche. Mi pare una questione di non poca importanza e quindi riteniamo che su di essa debba debba essere svolto il necessario approfondimento, non l'azione di disturbo che viene fatta da parte del senatore Furio Colombo, che vuole intervenire con argomenti estranei che appartengono al dibattito politico e non alla questione che stiamo affrontando.

anche perché lei ha dato la parola giustamente al senatore Furio Colombo. Senatore Colombo, abbia la compiacenza di ascoltare anche chi si rivolge a lei. Democratico senatore Colombo, non litighi col senatore Boccia, ascolti anche chi vuole rispondere alle sue cortesissime argomentazioni. sfoggio di grande cultura, io sono un uomo della strada e quindi non ho la possibilità di leggere quell'importante quotidiano. La invito, però, a vedere i siti Internet: troverà tantissima gioia espressa dal popolo italiano per la lezione che avete subìto nella giornata di ieri, perché quel giornale statunitense ha semplicemente registrato che siete andati ovunque a raccontare che avevate una maggioranza sulla politica estera e vi ha giustamente sbeffeggiato. Purtroppo, quel giornale non pubblica le foto dell'aggressione al senatore Rossi, che davvero vi avrebbero fatto vergognare per quello che avete combinato in quest'Aula. nuova finestra"). Vorrei invitare i colleghi, essendo in dichiarazione di voto su un emendamento, ad attenersi ai temi piuttosto rilevanti che hanno proposto il senatore Cantoni e il senatore Eufemi.

da parte di tutti oppure, se interventi provocatori vengono fatti, non può esserci negato il diritto di rispondere. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e LNP).* Vorrei ricordare al senatore Colombo che, ahimè, di scene scomposte quest'Aula è stata prodiga anche nel passato. Certo, la foto sull'«Herald Tribune» può non essere stata molto bella, ma ancora meno bella sarebbe stata una foto scattata verso l'altro lato dell'emiciclo, dove alcuni parlamentari a lei vicini, senatore Colombo, tentavano di impedire, con insulti, minacce e violenza fisica l'esercizio del diritto di voto da parte di un senatorie Va bene così, senatore Buttiglione, rivolgano una lettera al popolo italiano, perché non sanno qual è la politica estera del Governo, è un fenomeno inusuale, irrituale... PRESIDENTE. Va bene così, senatore Buttiglione, sono costretto a toglierle la parola; si attenga perlomeno al tema in discussione. Faccio un appello ai colleghi. Ovviamente ogni collega è libero di svolgere le considerazioni politiche e di merito che intende fare e io non posso impedire, senatore Buttiglione, Buttiglione, alcunché ai senatori che chiedono la parola. A norma di Regolamento, però, posso impedire che essi trattino materie che sono radicalmente estranee all'oggetto della nostra discussione. Questo lo posso fare.

Signor Presidente, desidero accogliere l'invito che lei ha rivolto ora all'Assemblea e quindi rinuncio al mio intervento,

che avrà letto, le dichiarazioni rese dal senatore Garraffa durante la seduta di ieri, come sono state tradotte quelle della Capogruppo dei Verdi

per invitarli a verificare le tecniche «pianistiche» che vengono adottate in questo emiciclo. Non vorrei,

«il contenimento dei costi a carico della clientela». È noto che il sistema bancario ha dei profitti notevolissimi, a livelli *record* mondiali, quindi non riusciamo a comprendere come non si sia ritenuto possibile tenere in considerazione un emendamento estremamente saggio, dove si invita al contenimento dei costi a carico della clientela. Vogliamo denunciare questo aspetto, che tiene conto di una impossibile correttezza per le aziende, soprattutto piccole e medie, che dovranno sopportare un notevolissimo costo, costo, ribaltato dal sistema bancario direttamente su di loro. Quando il relatore o il Sottosegretario daranno una giustificazione plausibile su questo emendamento logico e saggio ci adegueremo, ma siamo veramente in una condizione di grande imbarazzo.

di modificare questo decreto, e tra le questioni che ci parevano di un qualche interesse vi era anche quella del contenimento dei costi per la clientela. Questo perché? Perché noi vogliamo smascherare la demagogia della sinistra. rispetto ai grandissimi profitti, profitti *record*, realizzati dalle banche in questi ultimi anni, anche in una fase di basso profilo di crescita dell'economia, il il dito della sinistra si è appuntato contro il sistema bancario e poi, nel momento in cui c'è da affrontare concretamente una questione che riguarda clienti che possono essere imprenditori, piccoli imprenditori, assistiamo ad un atteggiamento di totale chiusura. Non basta sbandierare l'atteggiamento favorevole rispetto alla *class action*, alla tutela dei risparmiatori e a quanto è avvenuto con le vicende del risparmio nel nostro Paese se poi

Signor Presidente, in sede di dichiarazione di voto i Gruppi possono motivare politicamente l'espressione del loro voto. Allora, nell'associarmi a quanto detto dai senatori dell'opposizione, vorrei chiedermi come prenderà la stampa internazionale questo tipo di emendamento o la sua reiezione. Vorrei evidenziare un fatto, e su questo la prego di fare molta attenzione. So che questa mattina è stato approvato il processo verbale e quindi non si può tornare sul tema, però, evidentemente, c'è una distorsione mediatica del nostro dibattito. Leggerò semplicemente una frase del Resoconto stenografico della seduta di ieri, perché voglio immaginare che oggi vi possa essere lo stesso clima di ieri in quest'Aula: cioè ieri avremmo potuto approvare il decreto.

scendono verso il centro dell'emiciclo e inveiscono contro il senatore Zanone». Si registra questo dato. Successivamente, è scritto: «Il senatore Viespoli si avvicina al banco della Presidenza per fare una segnalazione». Ora, non sull'*«*Herald Tribune*»*, ma su tutti i giornali italiani abbiamo letto che vi sono state invettive anche contro il senatore Rossi, ma nel Resoconto stenografico non risultano. Vorrei dire a chi solleva certi problemi di fare bene attenzione a portare qui in Aula argomenti che non c'entrano nulla, e ribadisco: c'è stata solo arroganza nei confronti del senatore Rossi!

al sistema finanziario e bancario di applicare dei costi; diamo allora un timbro parlamentare anche alle liberalità e alle libertà di incidere su costi notevolissimi per la clientela, soprattutto delle piccole e medie imprese e delle famiglie.

della seduta odierna, perché i piccoli e i medi imprenditori dovranno avere la percezione che la sinistra è insieme alle banche.

a dimostrazione della confusione legislativa che regna in questo Governo. Abbiamo sottolineato altresì la necessità che la normativa contenuta nell'articolo avesse una basa omogenea.

presente, di intervenire per correggerlo, ma il diniego del Governo e della maggioranza è stato assoluto. Non possiamo però consentire che vi sia l'avallo

sulla direttiva MiFID e sulle fiduciarie - che tenga conto dei pareri espressi dalle Commissioni riunite nelle scorso mese di novembre sulla riforma del risparmio. Abbiamo assistito a tutto, anche all'aberrazione dello stravolgimento del progetto delle*Authority*, cancellato dal ministro Bersani, in difformità a quanto, invece, aveva fatto deliberare in quest'Aula dal vice ministro Pinza; stravolgimento degli assetti complessivi delle *Authority*. Naturalmente prendiamo atto che la maggioranza procede a sussulti e, quindi, non ci facciamo illusioni rispetto alla

riteniamo molto grave la decisione di approvare questa norma così come è stata portata in Aula. Mi associo alle considerazioni del collega Eufemi

noi rifiutiamo la logica di intervenire con gli ordini del giorno su norme sostanziali. Presidente Manzella, mi appello alla sua sensibilità:

C'è una gerarchia delle fonti che va rispettata, quindi rifiutiamo questo modo di procedere e di intervenire attraverso un ordine del giorno che impegni il Governo a tener conto del coordinamento legislativo. Se il coordinamento era necessario, andava fatto nell'altro ramo del Parlamento, dove sono stati compiuti errori. Pertanto, stiamo procedendo in modo innaturale, presidente Manzella. Mi rivolgo a lei e alla sua sensibilità; lei è un grande esperto di materia costituzionale e di diritto parlamentare: noi non possiamo procedere con questo metodo.

Presidente, intervengo su questo emendamento perché vorrei far sapere all'Assemblea che esso tenta di evitare una procedura di infrazione della Comunità Europea datata 1994.

Nessuno naturalmente mette in dubbio la buona fede del nostro ministro Alfonso Pecoraro Scanio, noto per essere contro la caccia, ma - a mio giudizio - risulta necessario ripristinare il ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio e la condivisione delle responsabilità di vigilanza del Ministero dell'agricoltura con le Regioni, per continuare ad assicurare, cari colleghi, il corretto bilanciamento tra la componente venatoria e quella ambientalista, nell'interesse generale della tutela dell'ambiente, e della corretta gestione agricola del territorio e nel più ampio rispetto dei concetti di ruralità e di biodiversità.

Il decreto presidenziale già prevedeva espressamente che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si adeguassero, nello stabilire le misure di protezione dei siti di Rete Natura 2000 (i cosiddetti SIC e ZPS), linee guida di carattere generale da adottarsi da parte del Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. autonome. Signor Presidente, capisco che questi possono essere argomenti di poco interesse, però inviterei i colleghi a riflettere, perché il mondo venatorio è rappresentato da 800.000 cacciatori. Come ho già detto ieri in quest'Aula, in discussione generale, vorremmo evitare che in questa assise si venisse a creare anche un movimento di cacciatori, oltre a tutti i movimenti che già ci sono. In questo modo, Presidente, si stravolge il testo del decreto presidenziale n. 357: si intendono annullare le linee guida già elaborate dalla LIPU e dal Ministero dell'ambiente, formalmente adottate con decreto ministeriale, in conformità ad un parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome e a vanificare l'operato normativo e regolamentare di quelle Regioni e Province autonome che, nel frattempo, hanno già provveduto a dettare disposizioni in materia, con riferimento ai principi indicati dalle predette linee guida.

ma dopo aver dovuto sostenere i 1.367 commi della legge finanziaria, che - come è stato ampiamente dimostrato non solo in quest'Aula, ma nelle settimane scorse

non istituisce strumenti adeguati alle esigenze dei nostri giovani, ma assegna un puro potere ed una disponibilità finanziaria ad uno specifico Ministro.

Con un Governo dimissionario, infatti, si vuole procedere con decretazione d'urgenza, al limite del tempo scadente, a regalare ad un Ministro dimissionario una vera e propria marchetta.

c'è una grande divisione sui princìpi generali che toccano la politica estera, ma c'è molta unità dove c'è ciccia da spartire. Nel caso specifico, la ciccia da spartire è conferire al fino ad oggi inutile Ministro con delega per i giovani un minimo di struttura da condividere con il collega Ministro per la solidarietà sociale, il quale fino ad oggi ha svolto il ruolo di sentinella di un partito nel Governo, ma poco ha contato nell'attuazione concreta. Il motivo grave per cui sono favorevole alla soppressione di questi articoli è che la costituzione dell'Agenzia comporta oneri rilevanti che sono destinati ad assunzioni di personale in aggiramento e in deroga alle norme generali previste nella legge finanziaria. Si tratta di un trucco di natura contabile che pesa non poco sul bilancio dello Stato creare letteralmente un minimo di struttura di propaganda ad un Ministro o a due Ministri che oggi ne sono privi. Non mi pare che Quintino Sella avrebbe approvato e non mi pare che il ministro Padoa-Schioppa non si trovi in un qualche imbarazzo, dato che ci sta dicendo che potrà ridurre le tasse solo dopo il 2009. Credo che, procedendo con norme di questo tipo, in cui si utilizzano disposizioni europee per aggirare la legge finanziaria e per provocare qualche piccola emorragia nel bilancio dello Stato, la riduzione delle tasse ce la sogniamo, salvo che prossime elezioni (io spero molto prossime, signor Presidente) non cambino i nostri ruoli in quest'Aula.

dal punto di vista economico e quindi del vincolo del bilancio e del risanamento, come pure sul tema affrontato la settimana scorsa

di natura costituzionale, con la crisi in atto, dovrebbero indurre ad un ripensamento rispetto all'urgenza di questa norma. Stiamo parlando di 13 unità con conseguenti oneri per consulenze e di due unità a tempo pieno; non sappiamo neppure che cosa avverrà rispetto alla definizione del nuovo Governo. Alla luce di ciò, abbiamo espresso delle preoccupazioni:

i cattivi maestri non possano trovare albergo nelle istituzioni; qui c'è bisogno di una presa di posizione ferma e io richiamo l'attenzione dell'Assemblea su questo punto.

Parlo adesso perché è stata addotta una serie di argomentazioni a favore della soppressione dell'articolo 5 che chiamano in causa argomenti che non fanno parte di questo testo e che solo

istituita in seguito a una decisione del Parlamento europeo e viene a sostituire e ad assumere le funzioni già svolte dall'Agenzia nazionale italiana della gioventù, che già esiste. C'è una risistemazione delle funzioni rivolte a promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, a sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza tra i giovani, in particolare per rafforzare la coesione sociale dell'Unione Europea, favorire la comprensione tra i giovani dei diversi Paesi, per contribuire allo sviluppo di qualità dei sistemi di sostegno alle attività dei giovani. Si tratta di una serie di misure tese a promuovere l'attività

Quanto poi all'accusa del senatore Baldassarri di una norma addirittura *ad personam*, mi pare che ci troviamo ad un'operazione di strumentalità senza limiti. Se volete sostenere che un'attività di cooperazione a livello europeo, cui l'Italia partecipi in modo organizzato con le politiche giovanili, è cosa inutile e dannosa ditelo con chiarezza, ma non affermate che la creazione

riferibili né in assoluto, né nello specifico all'articolo 5 le considerazioni fatte a proposito delle generazioni. Ora, dubito che

del ministro Ferrero, che non sappiamo se sarà ancora e nuovamente Ministro delle politiche sociali, sia rispettato tale principio di parità. Per queste ragioni, Presidente, invito ad un atto di coerenza tutti i colleghi che in passato hanno richiamato questa stessa

un'autentica espressione del mondo giovanile, questa è l'occasione per essere coerenti. Naturalmente, non ci facciamo illusioni sulla

di cui non è chiaro quanta parte della cifra indicata risulti essere già scontata nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio a legislazione vigente e quanta invece sia pienamente riconducibile alle esigenze conseguenti alla creazione di questa nuova struttura. Inoltre, si introducono elementi di rigidità nella tabella C, perché la metà del totale di detti oneri sembra caratterizzata da elementi notevoli di rigidità, trattandosi di spese di personale. Ora, abbiamo sentito la grancassa suonata nei giorni scorsi dal ministro dell'economia Padoa-Schioppa, che vuole riformare il bilancio,

rispetto alle decisioni che stiamo per assumere e sulle quali invito l'Assemblea a riflettere, per evitare, per così dire, di andare verso una deriva che porta all'annullamento del concetto concetto di verifica da parte dei nostri servizi e dei nostri uffici e quindi implicitamente da parte del Parlamento, che diviene esclusivamente luogo di ratifica di decisioni prese in altra sede.

ci troviamo di fronte ad argomenti che possono essere anche condivisibili ma che vengono blindati per l'inettitudine ad affrontarli nei tempi e nei modi opportuni, com'è successo con la legge finanziaria e con tanti altri provvedimenti in questi dieci mesi di legislatura; come è successo, invece, sotto altri

di voto favorevole, che voglio motivare richiamando tre articoli che ritengo importanti. Mi sarà concesso di richiamare l'articolo 4, perché interviene su una materia, sanando il mancato rispetto da parte di alcune Regioni della norma comunitaria in materia di specie cacciabili e di deroghe per quanto riguarda i calendari venatori. Sapete che l'Unione Europea è molto attenta a queste tematiche, quindi ritengo che c'era la necessità di intervenire anche attraverso l'emanazione di un decreto-legge. altrettanto positivo quanto previsto dall'articolo 5, perché istituisce l'Agenzia nazionale per i giovani, con relative risorse per le politiche giovanili.

di concessione del credito e quelli finalizzati a rendere più trasparenti i rapporti tra le imprese e gli istituti di credito. Valuto positivamente la modifica introdotta alla Camera secondo cui l'eventuale richiesta d'informazioni da parte delle imprese sul *rating* assegnato deve essere soddisfatta senza oneri a carico dei contribuenti; c'è la nuova disciplina del mercato e della trasparenza,

provocare alcuni problemi al nostro sistema economico e produttivo, formato prevalentemente da piccole e medie aziende. Tuttavia, credo sia una norma importante e ha fatto bene il Governo a intervenire attraverso l'emanazione del decreto‑legge.

Signor Presidente, non aggiungerò molto rispetto alle considerazioni che abbiamo svolto nella seduta di martedì e nel corso dell'esame degli emendamenti. Abbiamo sottolineato come questo decreto-legge sia uno coacervo di norme, cui si è aggiunta una sovrapposizione normativa con altre disposizioni comunitarie. Non è stata tenuta in considerazione alcuna proposta correttiva, neppure le indispensabili correzioni tecniche, come nel titolo, che è sbagliato nei contenuti.

e dalla necessità di adempiere ad alcuni obblighi comunitari in scadenza o già scaduti. Avevamo prospettato la soluzione di traslare

Se correzioni andavano fatte, esse andavano fatte in questa Camera, l'errore è stato commesso alla Camera dei deputati e lì, invece, si doveva intervenire. Noi ci siamo mossi, come UDC, con spirito costruttivo, soprattutto sulla direttiva di Basilea 2, proponendo miglioramenti e correzioni, dopo naturalmente quel lungo percorso elaborativo che c'è stato e che ha visto il coinvolgimento di tanti soggetti diversi, banche e imprese, stante le ricadute complessive sul versante del sistema. Riteniamo, però, che il Senato non possa essere solo il luogo della ratifica. Sottolineiamo - lo diciamo alla sinistra, che ha la stragrande presenza e maggioranza nella Conferenza delle Regioni - che anche sull'articolo 4 la Conferenza stessa aveva richiamato che la soluzione adottata non costituisca precedente, raccomandando invece un percorso istituzionale concordato. C'è poi questo capolavoro dell'articolo 5, che noi abbiamo richiamato, è un *cadeau* al ministro Ferrero; ritenevamo che in una situazione di crisi istituzionale, di Governo dimissionario, poteva essere evitato perché queste funzioni d'indirizzo delle politiche giovanili non avvengono a costo zero. Non abbiamo, tuttavia, sentito una voce da parte del Presidente della Commissione bilancio rispetto anche ai rilievi posti dal Servizio del bilancio. Tanto è vero che non è chiaro quanta stima della spesa è già scontata e quanta invece sia pienamente riconducibile alle esigenze conseguenti alla creazione della nuova struttura. E troppo generico è il vincolo all'utilizzo delle risorse conseguenti ai nuovi oneri per il personale. Avevamo presentato pochissimi emendamenti e, soprattutto su tale questione - lo ribadiamo - abbiamo sostenuto l'esigenza che fossero utilizzati giovani sotto i trenta anni, quelli nati dopo il 1977, dopo la contestazione di Lama, della quale ricorre quest'anno l'anniversario, e non i cattivi maestri della stagione degli anni di piombo. Veniamo a Basilea 2; la direttiva guarda alla stabilità del settore bancario, generando un forte legame tra banche e imprese. Cambiano i ruoli delle banche, siano esse grandi, siano esse medio-piccole, perché focalizzate appunto nella concessione di crediti alle piccole e medie imprese, valorizzando il localismo, dando attuazione ai principi di proporzionalità in relazione alle dimensioni, alle caratteristiche e alla rilevanza dei rischi. È un sistema di regole, appunto modulari, nella misurazione e nella gestione dei rischi. Le più forti preoccupazioni della nostra parte politica erano appunto per il sistema delle piccole e medie imprese e, soprattutto, le piccole e medie imprese italiane, come quelle tedesche, che hanno svolto analoga motivazione in sede comunitaria; perché le piccole e medie imprese hanno la caratteristica della impresa familiare, familiare, della bassa capitalizzazione e dei pluriaffidamenti bancari a breve. Allora, sarà necessaria una ripartizione della funzione finanza all'interno delle imprese e la qualità del rapporto banca-impresa assumerà maggiore rilevanza. Tuttavia, abbiamo posto anche un'altra questione che riteniamo è il problema della definizione della tassazione delle imprese bancarie, soprattutto delle obbligazioni che rappresentano un sostegno al finanziamento delle piccole e medie imprese. Speriamo

proclama pronunciato per compiacersi in qualche ambiente o con la sua maggioranza. Noi riteniamo che si debba procedere in questa direzione,

Grazie Signor Presidente, nel corso della discussione generale, il Gruppo di Alleanza Nazionale ha già avuto modo ed occasione di esprimere i rilievi e le perplessità

quanto è avvenuto nei giorni scorsi in Commissione finanze e quanto sta accadendo oggi in quest'Aula, perché non si è data all'opposizione la possibilità di aprire un franco dibattito. Ci si è sostanzialmente irrigiditi nel mantenere ferma la propria posizione, nonostante i fatti di ieri avrebbero dovuto determinare, all'interno della maggioranza e del Governo, una diversa disponibilità a dialogare con l'opposizione.

Recepire i regolamenti comunitari è assolutamente obbligatorio, perché è caratteristica dei regolamenti creare le condizioni e i presupposti per uniformare le normative degli Stati membri a quelli dell'Unione europea. Non è la stessa cosa, invece, per le direttive, che possono creare le condizioni per graduali riavvicinamenti tra le varie normative, ma devono tener conto, e non possono farne a meno, delle specificità nazionali. anche un altro problema, sempre di metodo: la cosiddetta disomogeneità della materia. All'interno di questo provvedimento, infatti, coesistono situazioni e questioni completamente differenti

linea di quanto si sta determinando già nel corso di questi anni all'interno dei Ministeri, dove avete creato le condizioni per un sostanziale *spoils system*, adottato in dispregio delle regole più elementari della difesa della dignità dei lavoratori. Lo avete fatto e lo continuerete a fare, adottando un sistema da autentica epurazione, al quale oggi vorreste aggiungere quest'altra ciliegina, in modo da creare le condizioni per fornire ad un Ministro, che non ha i requisiti, il supporto per poter determinare una politica assolutamente devastante. Noi peraltro, ed io personalmente, nel corso della discussione generale, avuto occasione di dire che il problema occupazionale va affrontato oggi in maniera complessiva, tenendo conto che, se continua ad esistere - ed in effetti esiste - il problema della disoccupazione giovanile, è altrettanto vero che esiste una disoccupazione che non è più prevalentemente giovanile. In Italia ci sono fasce di trentenni e quarantenni sostanzialmente espulsi dai processi produttivi dei quali non si interessano questa maggioranza e questo Governo.

Poi siamo passati ad un altro argomento importante, importantissimo, che ha tenuto banco nel corso di queste discussioni. Ci riferiamo a Basilea 2 e sappiamo perfettamente i suoi principi ispiratori: creare le condizioni per fornire solidità al sistema bancario soprattutto dopo che nel 1974, anno in cui nacque il comitato di Basilea 2, 2, accadde un fatto eclatante: il fallimento della Bankhaus Herstatt. Da allora si pensò di regolamentare ancor meglio il sistema dell'accesso al credito. Il problema serio è che oggi, mentre le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari continuano ad essere tutelati, l'alea e il rischio vengono scaricati sul sistema economico del Paese e non so se questo Governo si è reso conto dei disastri che sicuramente si produrranno sul sistema delle piccole e medie imprese, che in Italia, ancor più che in altri paesi d'Europa - è questa la specificità nazionale - sicuramente soffriranno per l'introduzione di tale normativa.

della presenza a Roma di ben 400.000 imprese, ma al contempo puntava l'indice sull'eccesso di indebitamento del sistema, tanto è vero che la Confcommercio affermava a chiare lettere che così questo sistema non poteva e non può continuare. continuare. Una parte di quel sistema sarà messo in ginocchio dall'introduzione scriteriata e senza alcun principio di Basilea 2 e ve ne assumerete fino in fondo le responsabilità. Questo perché non avete creato le condizioni per verificare il motivo cui tali imprese (polverizzate, tipicamente a conduzione familiare e attinenti a settori a rischio, quale quello della contraffazione e della concorrenza dei Paesi dell'est ed asiatici nell'ambito del costo del lavoro) ad un certo momento non riusciranno a reggere. Un sistema di piccole e medie imprese caratterizzato da scarsa redditività, da un alto indebitamento, da un'obsolescenza strutturale e da una discrezionalità anche nella concessione del credito. Che cosa avremmo dovuto fare? Non avremmo dovuto recepire Basilea 2? Avremmo dovuto sicuramente farlo, creando però le condizioni perché all'interno del nostro sistema vi fossero i presupposti per favorire il processo di avvicinamento a Basilea 2, fornendo, ad esempio, condizioni per dare servizi reali tendenti alla modernizzazione strutturale delle imprese, per rendere effettiva l'applicazione dello sportello unico, per prevedere interventi a sostegno di prestiti e mutui finalizzati alla ricapitalizzazione delle aziende. Tutto questo non è assolutamente accaduto. Allora il domani non è sicuramente roseo. Ci saranno moltissime imprese che non potranno più accedere al credito; ci saranno moltissime imprese che dovranno chiudere i battenti, che non potranno più guardare al futuro. Oggi il sistema delle imprese in Italia è diviso sostanzialmente in tre tronconi: il primo è quello che non ha sostanzialmente bisogno delle banche per poter operare e su questo non ci dilunghiamo analizzare i motivi per i quali è indifferente rispetto al sostegno creditizio. C'è un altro segmento che è quello delle imprese sostanzialmente fuori mercato, che non potrebbero e non dovrebbero ottenere crediti in nessun modo perché si tratta di imprese marginali. C'è poi un terzo segmento, quello più ampio, che copre una fascia maggioritaria, sicuramente superiore al 60 per cento, costituito da imprese che sono ai limiti della inclusione nei processi produttivi oppure nella estromissione delle stesse. Questo segmento va aiutato, se vogliamo sostenere il sistema Paese; va tenuto in conto, se vogliamo creare le condizioni per la salvaguardia di settori importanti dell'economia italiana; va tutelato, se vogliamo creare le condizioni affinché segmenti occupazionali non lievitino ancor di più, in senso negativo. Tutto ciò non è stato fatto perché state agendo, così come avete agito ieri

saranno ancora sudditi in un Paese assolutamente antidemocratico, come abbiamo verificato nel disegno di legge

ha interrotto la mia dichiarazione di voto appena dopo che avevo incominciato a pronunciare poche parole, con le quali io, a nome del Gruppo Per le Autonomie che mi onoro di presiedere, ho solo approvato i principi generali della politica estera del Governo tracciati dal ministro D'Alema. Il Presidente emerito della Repubblica, così come ha riportato il Resoconto stenografico della seduta, ha dapprima gridato «Vergogna! Sempre contro gli Stati Uniti!», per poi continuare con «Viva le SS del Sud Tirolo!». Lo stesso Cossiga, a seguito della mia risposta, nella quale ribadivo la democraticità del popolo sudtirolese, che ha sempre ripudiato le dittature fascista e nazista, che hanno provocato il dramma delle opzioni, ha poi contrattaccato rimarcando, rimarcando, in un comunicato, che nella sostanza del mio discorso sentiva già - cito - «l'eco della politica del grande Reich nazista» per cento della popolazione sudtirolese aveva fatto la scelta del regime fascista». Sebbene le dichiarazioni del senatore a vita Cossiga non si prestino ad un ulteriore commento, ritengo che rasenti la genialità che dopo la prima frase della mia dichiarazione di voto, nella quale, ripeto, non avevo espresso altro che l'approvazione delle linee del Governo, Cossiga sostenga che nel mio discorso sentiva già l'eco della politica del grande Reich nazista, un'accusa gravissima, ingiustificata, che respingiamo con fermezza. Lascia inoltre amareggiati l'uso alquanto disinvolto che il senatore a vita fa della storia del Sud-Tirolo e del dramma che la popolazione ha dovuto subire e vivere a causa delle dittature nazista e fascista. Le cosiddette opzioni, volute da Hitler e Mussolini, sono state un accordo scellerato, fatto sopra la testa delle persone, che hanno dovuto subire profonde ferite e lacerazioni personali e familiari. Si trattava di un patto che ha costretto i sudtirolesi a decidere se rimanere in Italia, rinunciando alla loro identità, alla loro lingua, alla loro cultura e magari essere trasferiti in altre province d'Italia, o andare in Germania, lasciando tutti i loro beni. Una drammatica scelta, imposta dalle due dittature, che ha portato grande sofferenza e diviso tante famiglie. Se poi più dell'80 per cento dei sudtirolesi si vide costretto, vista la forte pressione e propaganda dei due regimi, ad emigrare a malincuore, lasciando la propria terra e la propria casa, i propri masi, non fu è questo il motivo per cui ho preso la parola - un riconoscimento del nazismo, ma una scelta obbligata per salvaguardare lingua e cultura dalla pulizia etnica, messa in atto dal fascismo, che aveva proibito l'uso della lingua tedesca, chiuso le scuole tedesche e addirittura interdetto l'insegnamento religioso nella madrelingua, licenziato o trasferito in altre province i pochissimi dipendenti pubblici, licenziato gli insegnanti di lingua tedesca e cercato di sradicare tutti gli usi e le tradizioni locali. tradizioni locali. Siamo stupiti, e con me anche tutti i sudtirolesi, per la presa di posizione del senatore Francesco Cossiga. Il presidente Cossiga è sempre stato un grande amico del Sud-Tirolo, ha lavorato bene con i parlamentari altoatesini ed è stato garante del rispetto degli interessi della nostra terra. Per questo suo impegno gli siamo grati e proprio per questo non riusciamo a comprendere come sia stata possibile questa inqualificabile e superficiale offesa. Infine, signor Presidente, ringraziando anche lei per l'opportunità di poter parlare, colgo l'occasione per ringraziare i tanti colleghi del Senato che, sia per iscritto che oralmente, mi hanno espresso la loro solidarietà. ringrazio, senatore Peterlini. Devo dirle sinceramente che non ero a conoscenza di questo incidente che c'è stato, del quale mi rammarico molto mi auguro e spero che questo sgradevole fatto possa essere rapidamente chiarito, non solo tra lei e il suo Gruppo, ma fra l'intera comunità

di esprimere, a nome del Senato, una parola per quanto accaduto qualche giorno fa nell'aula di giustizia di un tribunale della Repubblica. Mi riferisco a quell'immagine di una bambina vestita di rosso fotografata da un cellulare in una gabbia insieme alla madre imputata in quell'aula di giustizia. Io credo che il Senato della Repubblica debba rompere l'incredibile silenzio che intorno a questa vicenda si è determinato perché, al di là delle iniziative del Ministro della giustizia, ritengo che quella scena debba trovare il Senato della Repubblica capace di esprimere un grande sdegno in nome della civiltà minima, soprattutto quando si tratta di bambini.

per precisare, anche doverosamente, che il procuratore generale della Repubblica ha immediatamente affermato che sul fatto in questione c'è stata una palese carenza di organizzazione degli uffici che dovevano occuparsene e dei diretti responsabili e che il Ministro della giustizia ha correttamente, immediatamente e senza indugio dato disposizioni agli uffici competenti per avviare un'immediata indagine conoscitiva e per sanzionare, se del caso, i responsabili, ove avessero omesso l'applicazione di norme di legge. L'intervento di questo Gruppo, a mio nome, non è però soltanto per riferire ciò che già gli organi di stampa hanno affermato, ma per qualificare come assolutamente indecoroso lo scenario rappresentato da telegiornali e giornali, per rappresentare e confermare la scelta di questa maggioranza di aumentare i fondi per la giustizia anche per migliorare questa assurdità, ma soprattutto (insieme al collega che mi ha preceduto dell'opposizione, ma credo insieme a tutti i colleghi presenti e assenti in questo momento) per segnalare che il Senato non vuole che questo capiti mai più.

voluta - la collega Finocchiaro. Credo sia importante ricordarci che nel nostro Paese, pur esistendo una legge che prevede per le madri detenute gli arresti domiciliari, e quindi apposite abitazioni per le stesse, affinché i loro figli possano condurre con le loro madri una

che vivono nelle carceri. Credo sia necessario, anche in un momento difficile per la vita politica come questo, che tutti insieme prendiamo una posizione sul tema in questione e pretendiamo che le leggi che il nostro Paese civile si è dato vengano anche rispettate e attuate.

dell'assunzione di iniziative organizzative di Procura e Ministero. L'ho fatto come meridionale, perché vorrei ricordare a me stesso che è accaduto nella città di Napoli, quella che doveva diventare la città dei bambini, e soprattutto in un Mezzogiorno dove si continua a ripetere con una stanca retorica meridionalistica che i figli «so' piezz' e core». Quindi, quello che è accaduto, proprio perché è accaduto in un'aula di giustizia, e in quella città, capitale del Mezzogiorno, a maggior ragione merita una espressione di sdegno da parte del Senato della Repubblica.

questi bambini, a questa bambina e a sua madre il senso della solidarietà e della vicinanza del Senato della Repubblica. Sono molto d'accordo con quanto proposto da lei, senatore Viespoli, del Senato tutto della Repubblica. Non ci interessano, nell'affrontare questa questione, le distinzioni politiche esistenti tra di noi: mi ha fatto piacere che lei l'abbia sollevata e che la sua la sua sollecitazione sia stata raccolta dalle colleghe e dai colleghi che sono intervenuti. Il nostro senso di vicinanza va oltre e al di là, come lei giustamente ha detto, dell'intervento,

Grazie